Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 7 aprile, quindi fino alla settimana successiva a Pasqua. Oggi pomeriggio, con eventuale prosieguo domani mattina, saranno discussi il decreto-legge in materia di competenza di tribunali e corti d'assise, nonché la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sull'uranio impoverito. Le rimanenti sedute dell'Assemblea previste per questa settimana, inclusa quella dedicata al sindacato ispettivo, sono sconvocate al fine di consentire i lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge in materia di enti locali,

nella giornata di martedì 23 marzo, in una seduta unica con inizio alle ore 10,30 fino alla votazione finale del provvedimento, con sospensione dalle ore 14 alle ore 15. Per i rimanenti giorni della prossima settimana resta confermata la decisione di non tenere sedute d'Aula in vista delle elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo. L'Assemblea tornerà poi a riunirsi martedì 30 marzo, alle ore 16,30, per l'esame del decreto-legge concernente l'Agenzia dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Nel prosieguo di tale settimana che precede le festività pasquali, il calendario prevede inoltre l'esame di ratifiche di accordi internazionali - tra i quali la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di esseri umani mozioni in materia di prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione e di politica estera, nonché lo svolgimento della relazione sul disegno di legge di riforma della professione forense. Nella settimana successiva alle festività pasquali l'Assemblea sarà convocata mercoledì 7 aprile, alle ore 15, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e di interpellanze e interrogazioni.

ricordare alla Presidenza del Senato che il 25 febbraio scorso, durante la discussione del disegno di

delle procedure di gara e del valore economico delle singole commesse. Sono passati 20 giorni e nulla appare sul sito della Protezione civile.

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale;

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, generalmente, nello svolgere la relazione o al termine dei lavori, il relatore ha il piacere di ringraziare coloro che hanno collaborato

su questi adattamenti al testo base, avremmo realizzato una positiva collaborazione proveniente da molti contributi. Voglio darne atto in particolare al presidente della Commissione, senatore Berselli, al cui impulso si debbono alcune accelerazioni virtuose, al sottosegretario Caliendo, che è venuto incontro a molte mie e nostre indicazioni,

Ci siamo impegnati, con una valutazione politica e tecnica al tempo stesso, prendendo le mosse da un provvedimento che per una volta tanto ha visto tutti d'accordo sui requisiti di necessità e urgenza, perché su questi anche la Commissione affari costituzionali si è espressa positivamente, e poi nell'affrontare il testo. Per essere estremamente sintetici, il testo propostoci dal Governo si è mosso innanzi tutto per venire incontro ad un'esigenza contingente ma di grandissimo rilievo, che aveva suscitato fondate e vive preoccupazioni.

di cassazione si è rivelato esservi stato quello che possiamo tranquillamente e senza polemiche definire un errore di talune magistrature di merito, che si erano pronunciate su una competenza che la Corte di cassazione ha censurato, facendo rilevare che una più attenta lettura delle norme avrebbe dovuto evitare il radicarsi errato della competenza Qualcuno ha voluto anche giustificare questo tipo di errore sostenendo che anche gli avvocati non avevano sollevato eccezione, ma è stato ribattuto, credo non senza fondamento, che gli avvocati sono difensori delle parti e che possono avere degli interessi strategici processuali Grazie, se è vero che in calce alle annotazioni di taluni nostri codici commentati la competenza sbagliata era indicata né più né meno come quelle magistrature di merito avevano ritenuto di poter fare. Ma, al di là di questa retrospettiva, che tuttavia è giusto anche menzionare in introduzione del provvedimento, il Governo si è mosso per sopperire a questa emergenza che si è creata e quindi, attraendo le competenze

quei processi molto importanti che pendevano, soprattutto a carico di organizzazioni di stampo mafioso o comunque di delinquenza organizzata, ed anche ad evitare che la scadenza dei termini di custodia cautelare nei confronti di un rilevante numero di soggetti

distinguendo quei procedimenti nei quali, così come voi potete leggere nell'articolo 2, 2, sia già stata esercitata l'azione penale salvo che prima della suddetta data sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise. Quindi, è stata correttamente disciplinata la situazione transitoria nella quale molti importanti procedimenti potevano venirsi a trovare. Non solo: il Governo, con una scelta di politica legislativa e anche codicistica comunque interessante, da qualcuno criticata ma dai più comunque presa in seria e positiva considerazione, ha ritenuto di intervenire, soprattutto con l'articolo 1, definendo - non solo per la contingenza o per i casi specifici ma a regime - la ripartizione più chiara delle competenze per ipotesi delittuose tra tribunale ordinario in composizione collegiale e corte d'assise. Questa è la sostanza del provvedimento che il Governo sottopone alla nostra approvazione. Ne abbiamo discusso molto approfonditamente in Commissione giustizia e all'esito della discussione - cui, come ho detto all'inizio, senatori della maggioranza e senatori dell'opposizione hanno dato un qualificato e penetrante contributo

che avrebbe ripartito le competenze tra corte d'assise e tribunale ordinario in maniera esplicita, cioè elencando tutti i reati che avrebbero fatto parte delle competenze della corte d'assise

ad una elencazione assai prolissa in una forma francamente poco congruente con l'esposizione in codice di questa delicata materia,

Sottoposte queste ipotesi al dibattito della Commissione, siamo arrivati ad una soluzione che mi permetto di definire largamente condivisa. Comunque, saranno gli onorevoli senatori a dare conto delle posizioni dei vari Gruppi. Il risultato

Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto comprensivo «Nicola Pecorelli» di Pago del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino. A loro rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio.

signor Presidente, cercherò di parlare, sperando nell'attenzione di tutti, a proposito di provvedimenti che riguardano l'amministrazione della giustizia.

In tal caso il limite massimo edittale della pena resta fissato in 24 anni di reclusione, limite che - come ha evidenziato la Cassazione nella sentenza della I sezione del 21 gennaio 2010, n. 4964 - coincide con quello fissato - *quoad poenam* - per l'individuazione dei reati di competenza della corte d'assise, fissato nell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale, La Cassazione, con la sentenza citata, pronunziandosi in un conflitto di competenza sollevato dalla corte d'assise di Catania, cui gli atti processuali erano stati trasmessi dal tribunale ordinario di Catania, ha stabilito che il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi del comma 4 dell'articolo 416-*bis*, appartiene alla competenza della corte d'assise e non a quella del tribunale, qualora la consumazione del reato associativo (che ha carattere permanente) si sia protratta anche successivamente all'8 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. La Cassazione ha inoltre sottolineato come, in base all'articolo 15 del codice di procedura penale, risulta attratto nella competenza della corte d'assise anche l'eventuale procedimento per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa necessariamente connesso. Mettendo insieme i due principi enunciati dalla Cassazione, numerosi processi relativi ad associazioni di tipo mafioso in corso in fase dibattimentale dinanzi al tribunale, se relativi a reati consumati dopo l'entrata in vigore della legge Cirielli (compresa l'ipotesi della permanenza del reato), erano esposti al rischio di doversi interrompere in seguito alla deduzione dell'incompetenza per materia del tribunale e di dover quindi iniziare nuovamente dinanzi alla corte d'assise. Erano, inoltre, a rischio di regressione anche i processi in corso nei successivi gradi di giudizio, ossia in appello o in Cassazione, poiché l'incompetenza per materia del giudice può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ovviamente, all'azzeramento dei processi poteva conseguire la scarcerazione di imputati cui venivano contestati gravi delitti di mafia. Il procuratore nazionale antimafia ha gettato giustamente l'allarme e il Ministro della giustizia ha riconosciuto la necessità politica di un intervento, teso ad evitare «l'azzeramento di tantissimi processi (oltre 380) e la scarcerazione temuta di tanti detenuti». Per arginare questo rischio il Partito Democratico, fin dal 9 febbraio 2010, ha proposto decisivi emendamenti al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, sulla funzionalità del sistema giudiziario in corso di conversione al Senato, finalizzando peraltro l'intervento esclusivamente alla soluzione dell'emergenza, ossia alla restituzione alla competenza del tribunale ordinario del reato di promozione, costituzione e direzione di associazione mafiosa aggravata. Gli emendamenti, bocciati in Commissione, sono stati proposti nuovamente in Aula, poiché l'intervento predisposto dal Governo con il decreto-legge oggi in esame affrontava non solo la modifica dell'articolo 5 del codice di procedura penale al fine di restituire al tribunale la competenza in materia di associazione mafiosa anche aggravata, ma, anticipando norme contenute nel disegno di legge n. 1440 di riforma del codice di procedura penale, estendeva la competenza della corte d'assise ai reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, ossia a tutti i reati attribuiti alla competenza delle procure distrettuali; ciò senza che sussistessero i requisiti di necessità ed urgenza e fosse prevista una copertura finanziaria per i costi, necessariamente conseguenti alla dilatazione delle competenze della corte d'assise e alla necessità di risorse umane, strumentali e finanziarie non disponibili a legislazione vigente e a bilancio invariato. Gli emendamenti del Partito Democratico sono stati respinti dalla maggioranza (sia pure per pochi voti) oggi ci troviamo a riaffrontare un problema che avrebbe potuto trovare definizione già nel febbraio 2007, poiché il decreto-legge sulla funzionalità del sistema giudiziario - già approvato all'unanimità alla Camera - avrebbe potuto essere definito in tempi brevissimi anche in seconda lettura.

del decreto-legge è faticosamente ricostruibile ma, tenendo conto delle previsioni del disegno di legge n. l'intento del legislatore è stato quello non solo di restituire al tribunale ordinario i reati in materia di associazione mafiosa ma anche quello di trasferire alla corte d'assise la competenza per tutti i delitti, tentati o consumati, ossia di tutti i reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia in materia di criminalità organizzata e di terrorismo.

ha presentato l'emendamento 1.100 che mantiene alla corte d'assise la competenza *quoad poenam* per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, escludendo i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazione di tipo mafioso e i delitti in materia di stupefacenti, che avrebbero determinato sicuramente un ulteriore intralcio per l'attività dell'assise. l'emendamento del relatore prevede l'aggiunta all'articolo 5 della lettera d-*bis*) che attribuisce alla competenza della corte d'assise alcune categorie di reati: delitti consumati o tentati di cui all'articolo 416, sesto comma, in materia di traffico di essere umani, delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

- è stato confermato in audizione dall'avvocato Spigarelli - sottolineano la necessità di una riforma organica della giustizia e non di interventi estemporanei. Il passaggio alla corte d'assise, ampliandone la cognizione, comporta per gli avvocati un problema. Essi mettono in luce che si dimentica che la competenza va fissata anche in base a considerazioni pratiche come - ad esempio - la frequenza statistica del crimine, la maggiore professionalità richiesta nel giudicarla e la maggiore speditezza nel reprimerla.

dal più alto numero possibile di giudici che il sistema consente. Questo secondo gli avvocati determina un *vulnus* nel sistema stesso e non è ragionevole. Guardando alle singole fattispecie di nuova cognizione, sempre l'Avvocatura fa presente che deve essere censurato l'inserimento dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602. Per questi delitti, infatti, la legge 11 agosto 2003, n. 228, in tempi recenti aveva escluso la competenza della corte d'assise proprio ritenendo più opportuno che il loro accertamento fosse devoluto ad un organo composto interamente da giudici togati. Nello stesso senso si sono espressi il Consiglio superiore della magistratura, la Direzione nazionale antimafia e l'Associazione dei funzionari dell'amministrazione della giustizia. Il secondo problema è costituito dal meccanismo di individuazione del giudice superiore per i procedimenti connessi di competenza del tribunale, disciplinato dall'articolo 15 del codice di procedura penale. penale. Associato alla proposta di modifica dell'articolo 5, lettera d-*bis*), determina infatti la *vis* attrattiva di delitti meno gravi rispetto a delitti più gravi. Quindi, il problema che si è posto il Partito Democratico - e per questo è intervenuto con un subemendamento - è di introdurre una eccezione a tale meccanismo di trascinamento della corte d'assise, laddove si intenda conservare la competenza della stessa evitando - ad esempio - che l'associazione finalizzata all'immigrazione clandestina - reato meno grave - sposti la cognizione in assise del reato di associazione mafiosa che pure era stata restituita al tribunale.

Signor Presidente, condivido la relazione svolta dal senatore Benedetti Valentini

per porre rimedio non solo al problema scaturito dalla sentenza della Corte di cassazione con cui si attribuiva la competenza,

- volendo intervenire per riattribuire al tribunale la competenza per il reato di associazione mafiosa anche aggravata, dopo aver detto questo alla lettera

estendeva la competenza al tribunale dei reati comunque aggravati dalle modalità mafiose, oltre che la competenza per i reati di associazione mafiosa aggravata. Con questa prima soluzione si attribuiva alla competenza del tribunale anche l'omicidio aggravato dalla mafiosità,

dopo aver escluso la competenza della corte di assise, con quel "salvo" si riattribuiva alla stessa la competenza per il reato di associazione mafiosa aggravata. Il bisticcio era troppo macroscopico per cui bisognava intervenire. Il problema che ci siamo posti è si interviene correggendo il decreto-legge (sperando che, nel frattempo, non siano stati commessi dei guai), ma si interviene solamente inserendo tra le esclusioni l'associazione mafiosa aggravata dall'essere armata

La discussione in Commissione giustizia su queste due posizioni è stata ampia e tecnicamente importante. La soluzione conclusiva, che vede l'adesione del Gruppo dell'Italia dei Valori (tant'è che in Commissione abbiamo ritirato il nostro emendamento ritenendolo assorbito dalla proposta di modifica del relatore alla quale si è aggiunta la nostra firma), è che i reati riguardanti le aggressioni alla persona nelle forme più manifestamente gravi (ossia

riequilibrato il problema relativo all'associazione di stampo mafioso, anche in coerenza con il trattamento di l'associazione aggravata (il traffico di stupefacenti era già escluso dalla competenza della corte d'assise). Dunque, si è riequilibrato il problema della competenza riassegnando, così come era sino al 2005, la competenza del tribunale per l'associazione mafiosa aggravata dall'essere armata e si è estesa estesa quella della corte di assise per i reati che vedono l'uomo come soggetto di particolari e gravi ipotesi delittuose. quindi concordi con il relatore per la soluzione che è stata adottata, ma, così come ho fatto in una precedente occasione nei giorni scorsi, mi preme sottolineare un problema, e ne faccio carico a lei, signor Presidente, perché se ne faccia interprete.

che approdano in Commissione giustizia siano formulati senza errori. Non è possibile uno scadimento della produzione legislativa così marcato. Ci vuole più diligenza. Non è possibile veramente che si debba continuamente intervenire per modificare dei testi che non sono adeguati al livello di quelli che provengono dal Governo. La prego veramente di farsi interprete di questo nostro disagio nel dover correggere dei testi maldestri.

di legge di conversione del decreto-legge che modifica in sostanza il codice di procedura penale, o meglio, le competenze della corte d'assise.

giurisprudenziale rispetto alla competenza per determinate materie e per determinati reati.

Cosa prevede questo decreto, che noi condividiamo appieno? Tampona di fatto la situazione:

Il decreto, in ogni caso, fa salvi tutti quei procedimenti che in corte d'assise abbiano già visto aperto il dibattimento (mettiamo al riparo da rischi praticamente tutto) e conserva anche l'efficacia di tutti gli atti compiuti (pensiamo agli atti irripetibili: ne abbiamo discusso qualche seduta fa). pertanto, tutto quello che è *in itinere* e tutto quello che si deve salvare. va giudicato, pertanto, per quello che è. Mi pare che anche l'opposizione non intraveda in questo provvedimento nessun tipo di taglio, né protezionistico né giustizialistico. secondo noi, se serve un'ennesima riprova, questo Governo sta dimostrando che non è assolutamente dalla parte della mafia, che non estremamente tempestivo per combattere la mafia e non perdere strumenti per combatterla. Di più, esso interviene non con legge,

poterli ritrovare: magari si potrebbero scarcerare dei detenuti già condannati per reati di associazione di stampo mafioso. La massima celerità, in questo caso, è d'obbligo. Da parte nostra, pertanto, al di là dei commenti che potremmo fare, vi è soltanto il sostegno e l'invito alla speditezza massima per non perdere ulteriore tempo ed evitare che questa giusta sentenza della Corte di cassazione

senza l'assillo dei temi derivanti dalle agende del Presidente del Consiglio e dai suoi problemi giudiziari e per la possibilità di parlare di questioni tecniche, sulle quali possiamo essere d'accordo, parzialmente d'accordo o in disaccordo, ma in una dimensione di fisiologia di dibattito politico. Condivido anch'io (e non sprecherò, pertanto, molte parole su questo punto) un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento di cui oggi ci occupiamo e sulla tempestiva adozione di misure che, ove non adottate, avrebbero generato problemi di allarme sociale e problemi legati alla possibile scarcerazione di soggetti pericolosi. Tali problemi, invece, sono stati appunto evitati con l'adozione del decreto. Al di là dei profili di carattere tecnico sulla scelta tecnica da adottarsi (mi si passi il bisticcio), e dei quali discuteremo in sede di discussione degli emendamenti, la questione fondamentale, a proposito del provvedimento del quale oggi discutiamo, è quella relativa al giudizio in ordine alla dilatazione delle competenze della corte d'assise o, per essere più precisi, all'allargamento delle competenze della corte d'assise. Io desidero fare un brevissimo *excursus* storico sulla funzione e sulla natura della giuria popolare e del giudice non togato, per poi esprimere una valutazione sulle scelte fatte in questo provvedimento. Noi tutti sappiamo che la giuria, storicamente, è un'istituzione caratteristica del diritto del diritto dei Paesi di *common law* (Regno Unito e Stati Uniti d'America in primo luogo e poi Canada, Australia e tutti gli altri). In quei Paesi, però, la funzione della giuria è funzione ben distinta, tecnicamente, da quella del giudice. La giuria, sostanzialmente, dice sì o no, in punto di fatto, sulla responsabilità dell'imputato, laddove tutte le questioni tecniche, sia di qualificazione giuridica che di procedura penale, vengono risolte dal giudice. La giuria emette un verdetto, che non è e non deve essere motivato, e il giudice decide sul *quantum* della pena, dopo il verdetto, dovendo invece motivare la sua scelta e fornire un resoconto tecnico delle ragioni della sua decisione. Nei sistemi cosiddetti di *civil law*, quali il nostro (che, in realtà, è un sistema ibrido, ma non mi dilungo troppo su questo punto), la corte d'assise è un giudice ibrido, nel quale alla funzione tecnica dei giudici togati viene coniugata una funzione di saggezza popolare e di introduzione del buon senso collettivo nella decisione in ordine a taluni rari reati, nei quali è prevalente l'accertamento di fatto e minoritaria la sussistenza di questioni di diritto, perlomeno dal punto di vista dell'interpretazione della norma penale. Si tratta di categoria necessariamente residuale, ove si consideri che i giudici non togati hanno il medesimo potere dei giudici togati in ordine a tutte le decisioni. Questo fatto, naturalmente, in presenza di questioni ad alto tasso di complessità tecnica, rappresenta un serissimo problema.

l'ambito di competenza della corte d'assise, si viene a creare un problema le cui conseguenze sono difficilmente prevedibili (o forse facilmente prevedibili), tra cui intasamento di uffici giudiziari rischio di ripetizione di processi (è bene non dimenticare che il nostro ordinamento prevede che, in tutti i casi in cui venga a cambiare solo per uno dei membri del collegio il giudice collettivo che decide, il processo deve ricominciare da capo), con un evidente problema, se il giudice è individuale o composto da tre persone, che diventa gravissimo se il giudice, come nel caso della Corte d'assise, è composto da otto persone. Non a caso, infatti, nei maxiprocessi di criminalità organizzata, per evitare questo genere di rischi, vi è l'abitudine di predisporre un doppio collegio, in modo tale che i giudici supplenti siano presenti allo svolgimento del dibattimento pronti ad intervenire e ad evitare eventuali reiterazioni, catastrofiche dal punto di vista dei termini di custodia cautelare e in generale dell'allarme sociale che ne deriva. Tutte queste sommarie considerazioni per dire (vado a concludere):

per l'estensione delle competenze della corte d'assise che, se fatta al di fuori di una riflessione organica sulla distribuzione di competenze e sulla natura stessa del giudizio penale, può produrre molti più danni di quanti non tenda ad evitare.

signore e signori del Senato, appunterò la mia attenzione sull'articolo 2, cioè sull'aspetto più importante del provvedimento che dobbiamo oggi valutare, per esprimere alcune mie perplessità sul contenuto di questa norma che salva i processi in corso. Ora, noi sappiamo che l'articolo 25, comma primo, della Costituzione prevede che nessuno possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nel caso di specie, ragioni politiche di necessità e di grande urgenza hanno indotto il Governo, prima, e indurranno questo Senato a votare una norma presenta alcuni aspetti di assoluta perplessità in riferimento al testo della Costituzione che ho poc'anzi ricordato.

e quindi accade che con questo provvedimento si tolga agli imputati di associazione mafiosa aggravata il giudice naturale precostituito, vale a dire la corte d'assise, affidando piuttosto questa competenza al tribunale. non ho sentito i costituzionalisti - che molte volte si sono espressi sollevando perplessità legittime su molti testi alla nostra attenzione,

questa norma difficilmente arriverà in Corte costituzionale perché per poter accedere ad essa bisogna che vi sia un tribunale, un giudice che ritenga la questione rilevante e non manifestamente infondata, e i giudici dei tribunali faranno scudo ai loro errori e a quelli dei loro colleghi. Se poi qualcosa passerà in Corte costituzionale faccio un'altra previsione: la Corte costituzionale dirà che va bene così per salvare la faccia e la responsabilità dei magistrati che hanno sbagliato. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, replico brevemente e volentieri al dibattito che qui si è svolto e che in qualche misura ha riecheggiato quello che si è svolto in Commissione. Intanto mi verrebbe fatto di dire che, paradossalmente, non tutti i mali vengono per nuocere, se è vero che la sentenza della Cassazione, oltre ad aver messo a nudo un errore che rischiava di perpetuarsi in chissà quanti altri casi, esponendoci a pericoli quantitativamente e qualitativamente ancor maggiori, ci ha dato comunque l'occasione per un intervento di razionalizzazione che, facendo convergere virtuosamente più volontà, ci aiuta a dare una sistemazione logica e corretta ad una situazione che rischiava di pendere ulteriormente con danni ancor superiori. La soluzione verso la quale mi auguro ci stiamo avvicinando e che con qualche compiacimento ho visto sottolineata con favore da alcuni Gruppi - il senatore Li Gotti lo ha fatto esplicitamente, ma anche altri onorevoli colleghi lo hanno fatto in maniera più o meno manifesta ci dà proprio la possibilità di dare un senso logico all'articolo 1 e alla sua portata e di inquadrare bene la *ratio* anche dell'articolo 2. Il senatore Li Gotti ci ha fatto fare una riflessione: ci ha fatto notare che l'auspicio generale di ciascuno di noi promana è che si debba arrivare a testi nella loro formulazione definitiva, ma anche a testi di ingresso, senza errori, non voglio dire grammaticali, ma anche senza errori di coerenza intrinseca. Vede, senatore Vede, senatore Li Gotti, ieri, se non erro, è stata la giornata della celebrazione dello *slow*, della vita "lenta", che naturalmente non significa rimanere indolenti o pigri o sordi all'esigenza del tempo e dei tempi, ma privilegiare l'esigenza di riflettere, privilegiare il bene e il meglio che non il piuttosto e il subito.

nel formulare osservazioni e nel cercare di migliorare anche i provvedimenti si scontrano spesso con le perversioni della politica militante, non solo parlamentare, che vogliono il far presto e il fare comunque perché altrimenti dopo non si fa più o rischia di insabbiarsi un provvedimento, mentre si dice che l'opinione pubblica richiede oggi decisioni rapide, incalzanti, addirittura in tempo reale. Questi sono i tempi in cui i testi sono sostituiti dalle battute di agenzia, in cui c'incontriamo per i corridoi e pretendiamo che si risponda addirittura in tempo reale, senza aver avuto nemmeno il tempo di pensare a questa o a quella battuta. È la politica delle battute, dell'apparire anziché della sostanza. Chi di noi è senza peccato a questo riguardo scagli un sacco di pietre, non soltanto la prima. Per quanto mi riguarda, spesso rischio d'esser tacciato di essere conservatore a questo riguardo, e infatti lo sono, perché sono amante delle grandi riforme e non delle riforme di apparenza: ma questo vuole il tempo, senatore Li Gotti. Bisogna che c'impegniamo tutti per cercare di far sì che questo non accada.

che per sua natura non può essere convocato ad ogni piè sospinto, per ogni reato anche di scarso allarme sociale o di scarsa incidenza sull'opinione pubblica.

di rango quale egli è, non manca di sottolineare che in definitiva, con questo provvedimento, stiamo spostando in corso d'opera la competenza per certi reati e per certi processi

definisce la corte d'assise - sia per il numero dei componenti del collegio, sia perché ne vengono a far parte giudici popolari, espressione della volontà popolare e della sovranità democratica applicata al potere giudiziario

Caliendo si è soffermato su questo argomento con onestà culturale, spiegandoci le ragioni per le quali l'Esecutivo ha ritenuto comunque di procedere su questo piano, con argomentazioni credo degne di attenzione e probabilmente anche di consenso. In altre parole, penso di poter dire al senatore Longo - se mi permette - che il principio del giudice naturale

e di poter tranquillizzare l'opinione pubblica rispetto a questa lettura che se ne può dare. Concludendo, credo che - al di là del tecnicismo che può appassionare i membri delle Commissioni giustizia e affari costituzionali, o comunque noi che ci fregiamo del pomposo nome di giuristi - al resto dell'Assemblea, pur avvertita sull'argomento, interessi soprattutto capire che al termine del nostro lavoro abbiamo dato, per un verso, una risposta ad un'emergenza di cui giustamente e doverosamente il Governo si è fatto carico con urgenza,

si è posto un problema se intervenire o meno con un provvedimento che tenesse conto della necessità di evitare la scarcerazione di pericolosi criminali, con qualche strappo alla regola della precostituzione del giudice, come ha ricordato il senatore Longo. Il dibattito in Commissione ha tenuto conto della volontà del Governo già manifestata con il disegno di legge n. 1440, che è ancora in corso d'esame al Senato, di ampliare la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. Personalmente sono convinto che, ove vi fossero disponibilità finanziarie molto più consistenti, sarebbe opportuno ampliare tale partecipazione dei cittadini all'amministrazione della giustizia. Probabilmente, come ricordava oggi il senatore D'Ambrosio in Commissione, dovremmo rivedere anche i criteri di partecipazione dei cittadini, tenuto conto che oggi nel nostro Paese vi è piuttosto un problema di disoccupazione intellettuale derivante da un enorme numero di cittadini già in possesso di laurea. Probabilmente i titoli di partecipazione dovrebbero essere rivisti. Ma rispetto al decreto-legge, così come confezionato, ha ricordato il senatore Li Gotti, il Governo ha presentato un suo emendamento, emendative sono state presentate anche dalle opposizioni e dal relatore. Sulla base di una discussione, si è pervenuti ad individuare un

apre una nuova finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta emendativa 3.1. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

di un'interpretazione autentica che tocca l'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale e determina la possibilità di procedere all'integrazione dell'articolo 5, comma 1, L'emendamento 1.200 serve ad evitare che in una disciplina transitoria possano verificarsi dei problemi tenendo conto che molti reati di associazione mafiosa aggravata devono ritornare alla competenza del tribunale.

alla formula dell'elencazione analitica, ma troppo prolissa, che io stesso avevo profilato di quelli che potevano essere i titoli di reato di competenza della

corte d'assise, il Governo ne ha proposta un'altra, più efficace dal punto di vista sistematico e sulla quale abbiamo lavorato con introduzioni e sottrazioni di competenza.

tuttavia, poiché esso va a colpire, sacrificare e minacciare il bene fondamentale della persona, la sua libertà, sembra più propriamente attribuibile alla competenza della

che suscitano forte allarme sociale e che ineriscono al bene della libertà e dell'autodeterminazione della persona.

quelli che attengono alle minacce di tipo terroristico allo Stato e alla convivenza civile della comunità nazionale.

Agli onorevoli colleghi che fossero interessati e che hanno ascoltato prima il dibattito preciso che abbiamo tenuto d'occhio anche il principio della competenza tecnica privilegiata, cioè abbiamo ritenuto che sia più corretto spostare il baricentro sul tribunale ordinario per quei reati che per la loro configurazione postulano un esame

forse anche trasversalmente, in quest'Aula e comunque nel dibattito politico tra coloro che optano nettamente e direi quasi pregiudizialmente, filosoficamente, per ampliare comunque le competenze della corte d'assise, perché ritengono che il coinvolgimento dei giudici popolari sia un valore in sé da estendere, da applicare a quante più fattispecie possibili, chi invece ritiene, al contrario, che si debba tradizionalmente riservare alla corte d'assise il giudizio sulle fattispecie delittuose particolarissimamente allarmanti e che attengono appunto all'aggressione ai diritti fisici e morali della persona, mentre si debba riservare alla tecnicalità più consolidata, più confermata, il giudizio sugli altri tipi di reato ritenendoli più numerosi. Infine, abbiamo tenuto presenti le esigenze di carattere organizzativo,

perché lo scopo evidentemente è quello di far funzionare la giustizia e non quello di incepparla. Questo ha dato luogo alla formula, che ritengo equilibrata (e mi rallegro che parecchi lo abbiano riconosciuto), dell'emendamento 1.100. Ciò mi consente, onorevole Presidente, dopo essermi dilungato troppo, di risparmiare il tempo rispetto al parere da dare sugli emendamenti perché, apprezzando il lavoro e anche la *ratio* ispiratrice degli emendamenti che sono stati presentati, mi permetto di auspicare un voto unitario sull'emendamento 1.100 che abbiamo costruito insieme nelle settimane scorse.

l'obiezione che viene formulata dal Sottosegretario è valida, in quanto andremmo a creare una ferita ulteriore all'ordinamento. Egli ha definito asistematica una norma di questo genere ed effettivamente è tale perché andrebbe ad introdurre un'eccezione all'eccezione, discriminando nel trattamento processuale tra reato e reato concepito nello stesso articolo, il che darebbe luogo a pasticci interpretativi forse anche più preoccupanti. Se vi saranno reati associativi finalizzati a quei reati che abbiamo trasferito alla corte d'assise, ben potrà quest'ultima occuparsi anche di quei reati. Questa è la ragione per la quale pregherei

G1, a firma Li Gotti ed altri, l'auspicio in esso contenuto - di dedicare più mezzi, più risorse e più personale alle esigenze di cui ci stiamo occupando - non può che trovarci d'accordo.

è anch'essa recepibile con la sola osservazione, senatore Li Gotti e colleghi, che ormai con molte normative siamo intervenuti su questo versante: basterebbe pensare alle norme di incentivo verso le cosiddette sedi disagiate, che non sono disagiate *tout court*, ma sono semplicemente le sedi nelle quali mancano le domande di magistrati per esservi destinati, il che non è assolutamente la stessa cosa. Quindi il Governo

un danno per l'amministrazione della giustizia. Tutto questo non perché a noi interessa particolarmente non spostare in assise taluni titoli di reati, ma per la preoccupazione che la corte d'assise, che è un organismo che funziona, possa essere ingolfata nel suo lavoro.

gli altri reati connessi alla sola ipotesi di delitti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera *d-bis)*. Per il resto resterebbe tutto fermo.

Il relatore ha proposto una modifica della norma principale, ossia quella che fissa le generali competenze delle corti d'assise, in maniera tale da escludere in maniera chiara la competenza per fatti di mafia a fronte di un allargamento minimo a fatti che non incidono in maniera evidente sulla funzionalità dell'organismo.

il disegno di legge di conversione del decreto-legge sarebbe stato assolutamente non votabile per le lacune gravissime che conteneva.

alcuni problemi. Io stesso, allorquando si è stabilita la competenza esclusiva del tribunale di sorveglianza di Roma in materia di proroga di 41-*bis*, mi ero posto il problema dell'articolo 25 della Costituzione. Mi è stato detto che stavo sbagliando e allora ho voluto ripetere il medesimo errore: per questo mi sono astenuto dal sollevare il problema dell'articolo 25 della Costituzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento, che risolve un problema gravissimo. Erano 338 i processi a rischio di azzeramento, con conseguente scarcerazione di boss mafiosi detenuti nelle nostre carceri. Questo provvedimento, con una norma peraltro scritta in maniera ineccepibile e quindi di facile interpretazione, definisce un equilibrio tra le competenze per materia del tribunale e della corte d'assise sul quale - siamo certi - la giurisprudenza non potrà ulteriormente intervenire con interpretazioni difformi. Per questo motivo il nostro voto sarà favorevole.

Il decreto-legge in discussione è sicuramente da condividere nella parte in cui interviene per attribuire la competenza al tribunale in composizione collegiale dei procedimenti per associazione a delinquere di stampo mafioso anche nelle ipotesi aggravate; ipotesi in relazione alle quali, sulla base della precedente disciplina, la competenza avrebbe dovuto essere attribuita alla corte d'assise con l'effetto di determinare un rischio - come dicevo anche in discussione generale - di annullamento per numerosi processi di mafia già celebrati dinanzi a vari tribunali. La scelta di attribuire al tribunale e non alla corte d'assise la competenza in materia di associazione mafiosa appare però ragionevole non soltanto rispetto al rischio contingente che possano essere annullati i processi già celebrati, ma in via generale e a regime. Si tratta sempre di procedimenti complessi, spesso fondati su attività di intercettazione, sulla valutazione di dichiarazioni di collaboratori, su indagini tecniche che richiedono la soluzione di complesse questioni tecniche e procedurali, uno studio approfondito del materiale probatorio e un'attenta valutazione delle prove che rendono necessaria una particolare competenza ed esperienza dei giudici professionali. Per questo motivo abbiamo ritenuto poco coerente con questa condivisibile scelta di escludere tali reati dalla competenza della corte d'assise l'attribuzione in questa sede di alcuni reati alla competenza della suddetta corte, pur dando atto che il testo, rispetto a quello proposto dal decreto-legge originario, è stato notevolmente migliorato. Resta peraltro sempre il rischio della possibile connessione dei procedimenti per i reati attribuiti alla competenza della con procedimenti relativi ad associazioni di tipo mafioso quando si tratti di un'associazione che si dedichi a sequestri di persona, oppure a contrabbando di tabacchi, come accade tuttora per alcune realtà che operano in determinate regioni d'Italia, o anche al trasporto di cittadini stranieri o al traffico di esseri umani. Ciò potrebbe vanificare lo scopo principale del provvedimento, perché in questi casi, non essendo stato approvato il nostro subemendamento, la competenza a giudicare sul delitto di associazione di stampo mafioso sarebbe attribuita

se commesse con finalità di terrorismo possano essere attribuite alla competenza del giudice ordinario o alla corte d'assise a seconda dell'interpretazione che si dà (quindi bisogna risolvere alcuni problemi di carattere interpretativo) oltre la necessità di rafforzare i collegi di corte d'assise. A questo riguardo, vorrei infatti ricordare che i collegi sono composti da otto persone e vengono spesso duplicati perché, accanto ai magistrati titolari, siano essi togati o popolari, si nominano i supplenti per evitare che la corte d'assise si paralizzi nella sua attività per un qualsiasi inconveniente che possa colpire un giurato. Questa è la preoccupazione che abbiamo portato avanti e che concerne solo la funzionalità della giustizia, ma di base resta naturalmente la necessità di dare un voto positivo a un provvedimento che il Partito Democratico ha ampiamente auspicato dal punto di vista politico per evitare che i processi di mafia potessero essere messi in non cale e potessero essere scarcerati vari imputati di fatti gravi che si trovavano anche nella fase di condanne già

Presidente, nell'annunziare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà, essendo già stato detto tutto sul piano tecnico, mi limiterò soltanto a due telegrafiche considerazioni. Vorrei,

bensì, con grande senso di responsabilità, si è cercato di porre rimedio a una situazione decisamente emergenziale. Grazie anche al lavoro in Commissione - credo sia giusto e doveroso sottolineare un'estrema disponibilità da parte del Governo nell'accettare un testo che era la sintesi del lavoro svolto

un percorso virtuoso di riflessione sul ruolo della corte d'assise che ha visto esprimere posizioni diverse: chi vi parla vorrebbe vederla come giudice prevalente, ma c'è chi ritiene che non debba esserlo. Non vi è dubbio che è emerso un dato estremamente significativo: quando si parla di dignità della persona e di fatti gravi che riguardano la persona riteniamo che la partecipazione popolare espressa nella

Signor Presidente, questa proposta di inchiesta parlamentare non vuole costituire un nuovo capitolo della storia infinita delle Commissioni di inchiesta sull'uranio impoverito. Essa parte piuttosto dalle risultanze della precedente Commissione la quale, nella XV legislatura, ha in qualche modo portato a compimento i lavori avviati durante la XIV legislatura

tra la presenza dell'uranio impoverito e l'insorgenza di patologie oggetto d'indagine, ma che proprio per questo si rende necessario allargare il campo dell'inchiesta onde capire e definire la natura e l'origine di alcuni fenomeni morbosi e patologici capaci di mettere a rischio la vita e la salute del personale militare e civile operante nei territori segnati da conflitti armati o comunque vicini a basi militari. militari. Venuta meno la possibilità di ascrivere tutta una serie di sintomi e patologie ad un quadro clinico unitario fondato sull'ipotesi del danno da uranio impoverito, si rende oggi opportuno verificare disturbi ed eventuali rischi sulla base di un quadro clinico per così dire aperto, contrassegnato cioè dalla presenza di molteplici fattori tra loro interagenti, al fine di conseguire condizioni di maggiore sicurezza per il personale militare e le popolazioni civili e al fine di definire con maggiore chiarezza responsabilità e condizioni giuridiche aventi riflessi pratici in ambito normativo, assicurativo e risarcitorio. La Commissione difesa, nel corso dell'esame delle proposte avanzate dai senatori Casson e Balboni, Balboni, con un proficuo lavoro, per il quale ringrazio il Presidente della Commmissione e tutti i colleghi, ritenuto di elaborare e di approvare un testo unificato dei due documenti, testo unificato che è stato poi successivamente integrato attraverso il recepimento di alcune proposte emendative. Il testo che pertanto si sottopone all'Assemblea offre una sintesi non solo delle proposte dei senatori Casson e Balboni,

Il primo punto è che l'attività di inchiesta della costituenda Commissione si soffermi, in particolare, su disturbi, patologie e danni messi in relazione alle pratiche di vaccinazione e all'azione dei vaccini in determinati contesti, vista la sempre più accertata gravità del fenomeno. Il secondo punto è che il campo di indagine della costituenda Commissione comprenda anche, in modo esplicito, i danni e i rischi derivanti dalla presenza in ambito militare dell'amianto e del radon. danni e rischi che il Ministero della difesa non ha mai sottovalutato, anzi, ma che debbono essere oggetto di un'inchiesta e di una valutazione da parte del legislatore. La nocività dell'amianto non ha bisogno di essere commentata e la legge n. 257 del 1992 impone la cessazione dell'impiego di tale sostanza. Tra l'altro, il Ministero della difesa fa parte di un gruppo di lavoro presso l'INAIL che si propone di estendere al personale militare le condizioni di cui godono i lavoratori, dato che l'INAIL dispone di un fondo per le vittime dell'amianto. un gas radioattivo naturale, la cui presenza è in funzione della composizione della morfologia del terreno e dei suoi substrati; è un prodotto del decadimento radioattivo del radio, il quale, a sua volta, deriva dall'uranio. L'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il radon come cancerogeno di gruppo 1, ossia come sostanza per la quale vi è evidenza accertata di cancerogenità anche negli esseri umani, collocandola al secondo posto, come causa di tumori polmonari, dopo il fumo di tabacco. Solo con il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il legislatore ha imposto ai datori di lavoro l'obbligo di effettuare la misurazione della concentrazione di gas radioattivo. Nel 2007 l'Amministrazione militare ha avviato un'indagine presso gli enti e i reparti delle Forze armate per acquisire l'esigenza di monitoraggio del radon. Tale attività ha generato la richiesta di effettuare misurazioni di radon presso 38 siti. È quindi un problema che esiste, anche se, allo stato attuale, sembrano esservi solo un paio di azioni legali nei confronti delle Forze armate in merito alla questione del radon. Il terzo punto emerso nel dibattito in Commissione difesa è che la costituenda Commissione, una volta istituita, debba approfondire immediatamente la questione dei risarcimenti. Oggi si tende a riconoscere la causa di servizio anche senza il riconoscimento di una malattia, ma nella presunzione che questa vi sia: ciò è giusto, ma lascia anche margini di eccessiva discrezionalità o ambiguità. Occorre perciò migliorare il sistema risarcitorio in termini di chiarezza e trasparenza, semplificando la normativa in materia, adottando procedure oggettive e cercando di equiparare il trattamento riservato alle vittime di patologie varie al trattamento riservato alle vittime del dovere e del terrorismo. Il quarto punto, infine, è che la Commissione d'inchiesta, una volta istituita, si avvalga anche della collaborazione del Comitato per la prevenzione e il controllo delle malattie costituito nel gennaio 2008 dal Ministro della difesa, al fine di indagare sui casi di malattia che hanno colpito i militari in missione e sul territorio nazionale, tanto più che tale Comitato è composto da esperti delle diverse competenze scientifiche, segnalate dal CNR, dalle università e dalla sanità militare, e potrebbe quindi fornire un ottimo supporto al lavoro della Commissione. Il testo proposto dalla Commissione difesa all'attenzione dell'Aula

La Commissione si impegnerà, sempre sulla base dell'oggetto indicato nell'articolo 1, ad attuare l'indicazione contenuta nella relazione finale della Commissione omologa della XV legislatura per dare continuità al lavoro L'articolo 2 delinea la composizione della Commissione, che prevede 21 senatori nominati dal Presidente del Senato rispettando la proporzione tra i Gruppi parlamentari e, ovviamente, l'articolo 2 prevede che sia lo stesso Presidente del Senato a nominare il Presidente della Commissione tra i componenti della stessa, perché la nomina di un Presidente di Commissione da parte del Presidente del Senato dà al suddetto l'autorevolezza necessaria a guidare una Commissione di inchiesta. L'articolo 3 precisa i poteri e i limiti della Commissione, che sono quelli dell'autorità giudiziaria, mentre l'articolo 5 statuisce che l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno. Il successivo articolo 6 prende invece in considerazione la pubblicità dei lavori richiamando tutti i membri della Commissione alla riservatezza di rispetto del segreto per tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti,

L'articolo 7 stabilisce il termine massimo per la conclusione dei lavori fissandolo in due anni con decorrenza dall'insediamento della Commissione. L'articolo 8 fissa, infine, le spese per il funzionamento della Commissione. In sostanza, il relatore auspica che l'Assemblea voglia esprimersi positivamente sulla proposta in esame, perché

istituire una Commissione per dare un presidio di serietà e trasparenza nel dibattito sull'uranio impoverito.

Oggetto dell'indagine delle prime due Commissioni sono stati i casi di morte e le gravi patologie che hanno colpito un numero significativo di nostri militari dopo essere stati impegnati nelle missioni all'estero o nei poligoni di tiro, ovvero nei siti di stoccaggio di munizionamenti. In sintesi, si trattava di verificare i possibili effetti di contaminazione derivanti dall'uranio impoverito, utilizzato nelle corazze dei carri armati, nelle munizioni anticarro e in diversi tipi di proiettili, e di quella che è conosciuta come «sindrome dei Balcani», ossia quella lunga serie di malattie - per lo più linfomi di Hodgkin e altre forme cancerogene - che hanno colpito i soldati italiani al ritorno dalle missioni di pace internazionale. di inchiesta che l'Assemblea del Senato oggi si appresta ad istituire (devo rilevare, signor Presidente, con un discutibile ritardo, tenuto conto che la Commissione difesa ha licenziato questo provvedimento già quasi un anno fa), un anno fa), ha un campo d'indagine più ampio rispetto alle precedenti, perché si è inteso includere nell'osservazione altri fattori di rischio per la salute emersi nel frattempo: tra questi in primo luogo l'amianto, che per lungo tempo è stato presente negli ambienti di servizio delle nostre Forze armate, soprattutto nelle navi militari, causando a molti militari imbarcati patologie asbesto correlate. Il campo di indagine si sviluppa inoltre sui vaccini utilizzati sul nostro personale militare, in merito ai quali si ritiene opportuno verificare, come segnalano alcuni indicatori, se in determinate condizioni non possano costituire un fattore di rischio. Ciò perché, se associati all'azione di un contesto di forte tossicità, potrebbero arrecare anch'essi vari disturbi e patologie. In ogni caso, queste ulteriori direttrici di indagine si pongono esattamente sulla linea del lavoro svolto dalle precedenti Commissioni, soprattutto nella XV legislatura: lavoro con il quale la Commissione che oggi l'Aula è chiamata a istituire dovrebbe, a mio avviso, porsi in linea di continuità, dandone quindi seguito. Si tratta, dunque, di una precisa assunzione di responsabilità che il Parlamento intende assolvere per la terza legislatura consecutiva, su un tema particolarmente delicato per l'attività dei nostri connazionali in divisa. Infatti, se inviamo i nostri contingenti all'estero in diversi teatri operativi per contribuire alla stabilità e alla sicurezza delle aree di crisi, e con questo intendendo adempiere ad impegni internazionali assunti dal nostro Paese, alla base di tale scelta vi deve essere parimenti un'assunzione di responsabilità anche nei confronti degli uomini e delle donne che ubbidendo al mandato loro conferito dal Parlamento partono in missione. E questo, nel caso in discussione, si traduce nel continuare ad indagare sfruttando tutti i progressi della scienza medica e dei metodi di ricerca - le possibili cause di disturbi e patologie, approntando quindi i necessari mezzi di protezione possibili per i nostri militari. In questo quadro quindi va letto l'allargamento del campo d'indagine, che pur partendo in particolare dalle missioni internazionali, non poteva escludere altre situazioni di rischio per la salute, quali la sicurezza dei luoghi di lavoro dei militari, la questione appunto dell'amianto. Il tema di indagine è quindi estremamente importante e, ora, ancora più articolato. Da questo punto di vista, l'impegno che attende la Commissione non può che partire dalle conclusioni emerse nelle precedenti indagini. In sintesi, quel lavoro consegna all'istituenda Commissione alcuni precisi punti. Le attuali evidenze medico-scientifiche, la scienza, non possono stabilire un nesso di causalità diretta fra la presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di gravi patologie. E non si conosce se e in quale misura le patologie riscontrate nei militari non siano invece derivanti dall'azione concomitante di diverse tossicità, tra cui, ad esempio, quella delle cosiddette nanoparticelle; constatato, però, l'obiettivo reiterarsi - in misura significativa - di patologie legate almeno in parte ai contesti dei teatri di impiego in cui ha operato il personale militare, si ritiene che esista un criterio di probabilità, di un nesso tra i due fatti. Da ciò deriva, da una parte, che se non si può escludere tale nesso, è dovere delle istituzioni continuare a lavorare per erodere questo margine di incertezza e quindi continuare ad aggiornare lo stato della conoscenza. Allo stesso tempo, si tratta di operare affinché si faciliti, per le vittime delle patologie e per i loro familiari, l'accesso a tutti gli strumenti di indennizzo previsti dalla legislazione Non quindi un semplice segnale di attenzione, ma un'attività concreta finalizzata alla riduzione dei rischi. Segnalo, in particolare, un effetto positivo ottenuto dalla precedente Commissione di inchiesta. La relazione evidenzia infatti che tra i principali ostacoli incontrati nel lavoro di indagine vi è stata la difficoltà, se non l'impossibilità, di disporre di dati completi e attendibili sui casi delle patologie oggetto dell'inchiesta, sia in riferimento al personale militare che alle popolazioni civili interessate. Di conseguenza, la stessa Commissione ha promosso una sistematica raccolta dei dati acquisiti presso tutti i distretti e i centri sanitari militari. Inoltre, ha indicato come priorità - sempre per facilitare la raccolta dati - una procedura di registrazione su supporto magnetico della storia sanitaria di ciascun militare, al fine di poter ricostruire tutte le diagnosi, le terapie e le misure di profilassi di cui ogni singolo militare è stato oggetto durante il servizio. Ora, signor Presidente, si tratta di riprendere quel lavoro, verificando in prima istanza - io credo - le risultanze di quelle significative indicazioni, per meglio proseguire l'azione di indagine. *(Applausi

oggi - direi finalmente! - discutiamo dell'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare che indaghi sui casi di morte e gravi malattie di personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccate munizioni ad uranio impoverito. La Commissione si occuperà inoltre dei fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno sul personale militare e sulla popolazione civile, con particolare attinenza, oltre che all'utilizzo di uranio impoverito, anche all'impiego di radon ed amianto. Si tratta di studiare approfonditamente, in particolare, gli effetti dell'impiego di proiettili ad uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico. Infatti, il diritto al lavoro ed il diritto alla salute sanciti dalla Costituzione impegnano certamente tutti noi a fare in modo che essi siano completamente accessibili a tutti i lavoratori, considerando evidentemente tali anche quelli che svolgono la loro attività in ambito militare. Sappiamo che spetta alla società e alla sua rappresentanza istituzionale operare affinché ci si occupi della salute e della durata della vita di chi opera nei luoghi di lavoro e, quindi, anche nei luoghi di lavoro militare. Sappiamo che anche nel 2006 è stata istituita ed insediata dal Senato una Commissione d'inchiesta, allo scopo di indagare sui casi di morti e gravi malattie che avevano colpito il personale impiegato prevalentemente all'estero in missioni di pace. Diverse sono state le difficoltà che la Commissione allora istituita ha incontrato, dalla parzialità dei dati, difficilmente completi ed attendibili, alla difficoltà di un monitoraggio costante del fenomeno. Allora si rilevò la necessità di avere uno studio più completo e tempi più adeguati per poter ipotizzare conclusioni non contestabili tra causa ed effetto, cioè tra le patologie riscontrate e l'esposizione all'uranio impoverito ad altri fattori di rischio ad esso collegati. Era noto che dal 1996 al 2006, 312 erano stati i militari ammalati di tumore, di cui 77 morti tra quelli operanti nei Balcani, in Iraq, in Afghanistan e in Libano. I dati erano parziali - come ho detto - e non si è ritenuto di poter disporre di una sufficiente valutazione comparativa ed adeguata che consentisse di analizzare compiutamente il fenomeno. Si può comunque dire che nella precedente legislatura, passando dal nesso di causalità al criterio di probabilità, si è comunque data una risposta a favore delle vittime e delle loro famiglie, così come si è potuto verificare che non risultava traccia in Italia dell'utilizzo militare di uranio impoverito. Non è mai stata invece convincente la risposta in tal senso delle altre forze militari in campo. Da più parti si è poi ritenuto di dover studiare il combinato tra le nanoparticelle e la somministrazione di vaccini per chi si recava in zona di guerra, questione che certamente andava ulteriormente approfondita, tenendo inoltre conto delle condizioni immunodepressorie o di eventuali altri squilibri dei soggetti in esame, che potevano anche avere individualmente. Per queste considerazioni la Commissione istituita nella XV legislatura aveva chiesto più tempo a disposizione per poter approfondire il lavoro e estenderlo, con particolare riguardo alle popolazioni residenti, sia alle zone di guerra sia alle zone antistanti i poligoni di tiro. Ecco dunque la necessità assunta unitariamente in questa legislatura di istituire questa Commissione di inchiesta parlamentare, in modo che ci si dia un tempo più lungo - due anni - per meglio definire il quadro causa‑effetto tra gli agenti patogeni e l'eventuale insorgere delle patologie: non è detto che quanto non è stato trovato oggi non si possa trovare successivamente. Serve un'adeguata raccolta e un'analisi epidemiologica dei dati sanitari e relativi al personale militare e civile. Serve una nuova attenta analisi della composizione dei vaccini somministrati e delle modalità della loro somministrazione, nonché un più puntuale monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti vaccinati. Si coglie, inoltre, l'occasione dell'istituzione della Commissione per trattare gli effetti dell'esposizione dei militari, e non solo, anche al radon ed all'amianto, materiali per i quali è già assodata la natura patogena

verificati i luoghi di esposizione ed i rischi conseguenti per il personale militare e civile esposto. Va infine studiata la natura dell'indennizzo previdenziale ed il sostegno al reddito per i pazienti, le vittime e le loro famiglie. È inoltre scontato che in base al principio di precauzione sarebbe importante che il nostro Paese intervenga nelle sedi opportune perché l'uranio impoverito non sia più utilizzato a fini bellici, stante la sua natura radioattiva e genotossica ed i sicuri effetti di inquinamento ambientale, come già fortemente affermato dalla letteratura internazionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è per la terza legislatura consecutiva che il Parlamento procede all'istituzione di una Commissione di inchiesta sui casi di morte e sulle gravi patologie che hanno colpito un numero significativo di nostri militari.

diramò un documento contenente la descrizione dei rischi associati all'esposizione all'uranio impoverito. Nello stesso periodo, l'opinione pubblica venne a conoscenza di denunce in base alle quali si stava manifestando un consistente aumento dell'incidenza di gravi patologie, in particolare di neoplasie tra i militari che avevano preso parte alle missioni nei Balcani. Il Parlamento in quell'occasione fu tempestivo e decise di avviare un'attività conoscitiva al fine di approfondire una questione che stava assumendo connotati particolarmente allarmanti. I primi atti del Parlamento furono un'indagine conoscitiva della Camera dei deputati e poi la cosiddetta commissione Mandelli. Purtroppo questo pur considerevole sforzo non ha portato ad alcuna certezza né allora, né nelle Commissioni d'indagine successive. Mentre l'associazione Vittime Uranio, infatti denuncia 216 morti e oltre 2.500 malati, l'ultima Commissione parlamentare in materia, due anni fa è giunta a conclusioni molto più incerte. Essa, ha stabilito che allo stato delle attuali evidente medico-scientifiche non si può stabilire un nesso di causalità diretta fra la presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di gravi patologie. non si sa se ed in quale misura le patologie riscontrate nei militari non siano invece derivanti dall'azione concomitante di diverse tossicità. *(Brusìo).* Io capisco, signor Presidente, che ormai quest'Aula è appiattita è appiattita su decisioni che vengono prese in altre sedi, però un minimo di attenzione o almeno un minimo di rispetto per l'Aula stessa sarebbe auspicabile. Visto, Visto, tuttavia, il reiterarsi, in misura significativa, di patologie, legate almeno in parte ai contesti dei teatri operativi in cui ha operato il personale militare, la Commissione della XV legislatura ha rilevato l'esistenza di un criterio di probabilità nel collegamento tra i due fatti. Criterio di probabilità che impone alle istituzioni alcuni doverosi provvedimenti, tre in particolare. Occorre, anzitutto, apprestare tutte le possibili tutele previdenziali e amministrative ai militari ammalati e ai loro familiari. È indispensabile, poi, continuare a lavorare per erodere il margine di incertezza, approfondendo la nostra conoscenza in materia e aggiornando quanto più possibile i dati, ovviamente, è doveroso mettere a disposizione del personale tutte le protezioni possibili. Questi, onorevoli colleghi, sono oggi gli obiettivi della Commissione parlamentare che vogliamo istituire. Questo il senso della sua esistenza: capire cosa è accaduto sin qui, risarcendo vittime e familiari e lavorare perché non accada più, allargando quindi, rispetto al passato, l'orizzonte di riferimento. La Commissione che il Senato oggi si appresta a istituire ha un campo d'indagine più ampio, perché si è inteso includere nell'osservazione altri fattori di rischio per la salute che sono emersi nel frattempo. In particolare l'amianto, che per lungo tempo è stato presente negli ambienti di servizio dei militari, a cominciare dalle navi militari, dove un elevato numero di personale delle Forze armate ha contratto patologie asbesto-correlate. i vaccini, in merito ai quali si ritiene opportuno verificare, come segnalano alcuni indicatori, se in determinate condizioni non possano costituire un fattore di rischio per i militari. importante oggi sottolineare anche la funzione per così dire etica che deve rivestire la Commissione. Essa, infatti, deve anzitutto rappresentare la precisa assunzione di responsabilità che il Parlamento intende esprimere in questo delicato ambito per la terza legislatura consecutiva. In tutte le missioni all'estero esistono dei fattori di rischio; dovere improrogabile delle istituzioni, tuttavia, è eliminare i rischi calcolabili, ossia quelli che si possono circoscrivere ed eliminare, facendo il possibile per ottenere il massimo della tutela per le condizioni di salute dei militari. Questo si traduce nel continuare ad indagare tutte la cause di disturbi e patologie, mettendo nel contempo a disposizione dei militari tutti i mezzi di protezione possibili. Per questo abbiamo voluto ampliare il campo d'indagine della Commissione e portare all'attenzione del Parlamento, oltre alla particolare situazione delle missioni internazionali, anche il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro dei militari. L'orizzonte dell'indagine è quindi estremamente ampio. L'invito, non scontato, è di partire dai dati. Ad oggi non esiste un censimento completo ed aggiornato dei militari colpiti da patologie riconducibili alle cause di cui trattiamo e questo compromette l'attendibilità di ogni possibile conclusione o provvedimento in materia.

colleghi che hanno toccato le motivazioni che inducono il Senato a voler approvare la costituzione di questa Commissione d'inchiesta.

l'origine delle nanoparticelle dei metalli pesanti che non sono presenti in natura e che sono stati trovati nei tessuti dei militari italiani che si sono ammalati, molti

oltre a trovare le conferme in statistiche epidemiologiche, necessarie ad acclarare ulteriormente questo grave fenomeno che ha colpito

chiudere il cerchio, nel senso di trovare le motivazioni medico-scientifiche che dimostrino che l'assorbimento, anche in quantità notevoli, a livello cellulare delle nanoparticelle nei tessuti dei soldati ammalati abbia come conseguenza il crearsi di situazioni di un percorso che, a mio parere, deve essere scientificamente affrontato in maniera molto attendibile, anche se è complesso. Una delle difficoltà che abbiamo incontrato nella Commissione che ho presieduto è proprio quella delle dimensioni dei campioni epidemiologici a disposizione, che sono limitati rispetto alla scelta alla scelta comune di analisi epidemiologica di fenomeni come questo e che invece trovano, come è riportato anche nel testo della proposta di istituzione di questa Commissione, altrettanta difficoltà, ma per versi opposti, nell'individuare all'interno delle popolazioni civili

la distruzione fisica degli archivi sono elementi che causeranno delle difficoltà alla Commissione nell'individuare in una popolazione così ampia e variegata, che negli anni ha avuto delle migrazioni - ripeto - abbastanza consistenti, È importante comunque proseguire; è importante anche valutare le problematiche relative ai vaccini. La Commissione che ho presieduto non ha potuto sostanzialmente affrontare questo tipo di aspetto, che

per quanto riguarda l'aspetto del risarcimento dei danni, ma soprattutto per quanto riguarda le protezioni che i nostri soldati attualmente impegnati nelle missioni internazionali di pace hanno ovviamente diritto di avere avere a difesa della propria incolumità nel momento in cui operano successivamente ai bombardamenti che avvengono nei teatri bellici. Ma ciò è importante anche allo scopo di individuare delle motivazioni scientificamente avvalorate e acclarate sul fatto che la presenza di queste sostanze nel tessuto umano poi generi le neoplasie, i linfomi e le leucemie che abbiamo riscontrato.

ad uno scambio di opinioni con chi ha svolto nel tempo questo importantissimo lavoro, in modo da fornire nei tempi più rapidi possibili e con le misure più circostanziate possibili delle risposte ai soldati delle risposte ai soldati che sono impegnati attualmente nelle missioni internazionali e alle famiglie dei militari che invece hanno dovuto subire conseguenze importanti sul proprio fisico, o addirittura la morte per il servizio che hanno dato al nostro Paese.

e continuiamo a ritenere, che la loro vita e la loro salute debbano concretamente essere tutelate di fronte ai pericoli che quotidianamente essi sono costretti ad affrontare nell'esercizio delle loro funzioni. Per questo abbiamo assiduamente sostenuto, con estrema convinzione, la necessità di garantire ai nostri militari di stanza all'estero adeguate misure precauzionali, nonché efficaci equipaggiamenti di protezione individuale, al fine di di diminuire sensibilmente l'insorgere di gravi patologie tumorali e non, ed evitare quei danni morali e fisici destinati a segnare la vita dei nostri uomini una volta tornati a casa. È un dato di fatto ormai che decine di soldati siano tornati dalle missioni internazionali offesi da contaminazioni derivanti da contatto con l'uranio impoverito. Rispetto a questa tragica certezza, riteniamo che la politica non possa più far finta di niente e che lo Stato abbia il dovere di non abbandonare coloro che, spesso in giovane età, hanno deciso di lavorare all'estero per la Patria e, tornando, si trovano costretti ad affrontare malattie insidiose e spesso mortali, senza che venga loro riconosciuto alcun risarcimento. Cari colleghi, ritengo che questo sia il punto fondamentale su cui si deve intervenire. Non si possono più accettare atteggiamenti bifronte del Governo, della maggioranza e della politica rispetto a tale problema. Non si può più retoricamente inneggiare alla presenza dei nostri militari all'estero, colmandoli di lodi per i compiti che svolgono nei molteplici e difficili fronti su cui operano, e poi

sono impegnati, in contesti fortemente degradati dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario; contesti caratterizzati, soprattutto, dalla presenza di uranio impoverito e dalla dispersione delle cosiddette nanoparticelle, ossia polveri ultrasottili prodotte dall'esplosione di materiale bellico che, se inalate ed ingerite, producono gravi danni alla salute. Su questo aspetto il Parlamento ha istituito, già nella XIV e XV legislatura, un'apposita Commissione di inchiesta. Nonostante la desolante parzialità dei dati a disposizione, da quanto si evince dalla relazione finale dei lavori, l'ultima Commissione parlamentare di inchiesta, prendendo atto che i dati e le ricerche disponibili non confermavano, ma nemmeno escludevano, il possibile legame tra l'insorgere di patologie gravi tra i nostri militari e l'esposizione all'uranio impoverito o altri agenti nocivi da parte degli stessi, ha intelligentemente sostituito il nesso di causalità, impossibile da provare direttamente, con l'utilizzo di strumenti statistico-probabilistici. In base a tali strumenti si stabilì che il verificarsi dell'evento morboso su militari che abbiano operato in contesti fortemente degradati ed inquinati costituisce, a meno che l'amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità, elemento sufficiente a determinare, per le vittime delle patologie e per i loro familiari, il diritto a ricorrere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente. Oltre a tentare di chiarire tale aspetto, la suddetta Commissione sottolineò la necessità di disporre di un quadro più chiaro e preciso del numero di militari effettivamente contagiati. A tal proposito, nelle sedute del 9 ottobre e 6 dicembre 2007, il ministro Parisi fornì, per il periodo 1996-2006, dati già abbastanza significativi sui casi di malattia accertati e sui militari deceduti - rispettivamente 312 e 77 precisando che solamente per il quinquennio 2002-2006 esisteva una raccolta informatizzata da cui poter evincere il numero preciso di militari partecipanti alle missioni nei Balcani, Iraq, Afghanistan e Libano. Da tale raccolta risultarono 56.600 unità totali, di cui ben 216 si sarebbero ammalati di tumore. Nonostante i numeri ufficiali del Ministero, non posso però - cari colleghi - non tenere conto delle cifre che vengono invece fornite dall'Osservatorio militare, secondo cui, dagli anni Novanta ad oggi, i militari deceduti in seguito a patologie oncologiche sarebbero circa 170 e i malati più di 2.500. Si tratta di dati che dimostrano ulteriormente la pericolosità delle missioni internazionali che hanno visto, e vedono tuttora, impegnati i nostri militari. Anche per fare maggiore chiarezza su queste tragiche cifre venne istituito, il 23 novembre 2007, un apposito organismo di ricerca denominato «Comitato per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della difesa» che, composto da ricercatori di assoluta competenza scientifica, selezionati dai Ministeri della difesa, della salute e della ricerca, avrebbe dovuto assicurare una conoscenza e una valutazione più completa del fenomeno. Ben presto, però, di tale Comitato si sono perse le tracce e, a tal proposito, in data 25 settembre 2008, il collega Pegorer presentò in Commissione difesa un atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedeva se fossero emersi, nell'anno di attività dello stesso, elementi di novità rispetto alle conoscenze scientifiche ed alle conclusioni cui erano giunte le Commissioni parlamentari di inchiesta istituite nelle legislature precedenti. Rispondendo nella seduta del 28 ottobre 2008, il sottosegretario Cossiga precisava che la raccolta delle informazioni sanitarie e di impiego, fornite dagli Stati maggiori di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, relative al personale militare impiegato nei teatri operativi dei Balcani, del Libano, dell'Iraq e dell'Afghanistan, era in fase di affinamento conclusivo e che i dati erano in corso di elaborazione e valutazione presso l'Osservatorio epidemiologico militare, da tempo istituito presso la Direzione generale della Sanità militare. Tuttavia, cari colleghi, a distanza di un anno e mezzo non abbiamo ancora alcuna comunicazione in merito alla elaborazione dei suddetti dati, nonché delle risultanze da essi derivanti. Chiedo, pertanto, che si possa, nel più breve tempo possibile, accedere a notizie più precise al fine di verificare l'avvenuto svolgimento dell'attività di studio ed approfondimento per cui il Comitato è stato appositamente istituito. L'uranio impoverito e le nanoparticelle non sono, però, le uniche cause di gravi malattie per i nostri militari. A tal proposito, non possiamo essere indifferenti nei confronti dell'esposizione all'amianto che, negli ultimi dieci anni, ha stroncato la vita di oltre 300 militari imbarcati su navi imbottite di asbesto. L'amianto era presente in molte imbarcazioni della Marina militare, in particolare sia nei dragamine e cannoniere consegnate dalla Marina americana dopo la fine della seconda guerra mondiale e l'ingresso dell'Italia nella NATO, sia sulle navi costruite successivamente, tanto da doverle sottoporre, in tempi recenti, a bonifica. Macchinari, tubature, cabine: tutto era rivestito con il minerale tossico, in forma pura o impastato con altro materiale. Il quotidiano contatto con questo tipo di materiali fino al 2005, e cioè fino al disarmo definitivo, ha rappresentato una tomba silenziosa per molti nostri militari. Una convinzione, cari colleghi, provata dal fatto che lo scorso settembre il Ministero della difesa, primo e finora unico caso nella storia della Marina militare, ha risarcito con 850.000 euro (per ognuna) le famiglie di due marinai uccisi da mesotelioma pleurico, il tumore da esposizione all'amianto. Inoltre, tale risarcimento è arrivato a sorpresa, prima ancora che i giudici del tribunale di Padova si pronunciassero sulla richiesta di rinvio a giudizio, presentata dalla procura e successivamente accolta, per 14 ammiragli della Marina, indagati per omicidio colposo e inosservanza delle norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. In pratica, il Ministero della difesa ha pagato prima della sentenza, ammettendo di fatto che la morte dei marinai in questione fosse necessariamente da relazionarsi al contatto con le navi Tutto questo mentre giace da più di un anno in Commissione lavoro e previdenza sociale il disegno di legge, presentato dal collega senatore Casson, recante disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, con il quale si vorrebbe concretamente e ambiziosamente bonificare dalle migliaia di tonnellate di fibre di amianto e di cemento-amianto l'ambiente, gli edifici privati e pubblici, le fabbriche, nonché realizzare forme adeguate di tutela sanitaria e garantire l'efficiente funzionamento del Fondo per le vittime dell'amianto istituito con la legge finanziaria del 2008. A tal proposito, è di difficile comprensione la differenziazione in termini di trattamento risarcitorio per danni subiti da amianto tra le vittime civili e quelle militari. Ho fatto riferimento, in questo mio intervento, a fatti ben precisi perché ritengo che in relazione al documento in discussione oggi, finalizzato, sulla falsariga delle due precedenti legislature, alla istituzione di una nuova Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito, non si debba dimenticare il nostro vero obiettivo: la tutela della salute dei nostri militari, nonché il riconoscimento, in tempi brevi e non cadendo nella lentezza burocratica, degli eventuali danni subiti dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni. Credo infatti, esimi colleghi, che il messaggio che questo emiciclo ha il dovere di inviare ai soldati malati e alle loro famiglie debba essere anche di altra natura: chi ha messo a rischio la propria vita e la propria salute per la patria, al punto da ammalarsi seriamente, deve necessariamente poter contare sulla presenza dello Stato, deve poter fare affidamento su un sistema di aiuti economici ben definito e non farraginoso che gli permetta di curarsi nel miglior modo possibile. Su questo punto non possiamo più concederci alcuna minima esitazione. Mi auguro quindi, cari colleghi, che entro e non oltre la legislatura si giunga ad una soluzione chiara, definitiva e concreta di tale problema.

al quale voglio riconoscere il pregio di aver trattato la materia con equilibrio, con grande disponibilità alla comprensione e alla accettazione delle molteplici sensibilità rappresentate e al quale chiedo, se posso permettermi di farlo preventivamente (ma questa è l'unica sede che ci viene riconosciuta), l'eventuale disponibilità in sede di replica a confermare oppure smentire l'interpretazione che il nostro Gruppo dà ai molteplici valori fondanti che riteniamo di dover riconoscere nel provvedimento che stiamo esaminando.

un impegno morale che abbiamo ripetutamente assunto e che in ogni occasione utile confermiamo nei confronti dei soldati che vanno a rappresentare il nostro Paese nelle missioni di pace all'estero. Ad essi noi chiediamo di essere portatori dei valori

però un altro impegno che abbiamo assunto come parlamentari di questa Repubblica è quello di onorare l'articolo 32 della Costituzione, che parla non solo di diritto alla salute, ma sostiene l'inderogabilità rispetto al dovere verso la salute, verso la garanzia della salute. ragioni, i temi di cui stiamo parlando oggi si sviluppano, se possiamo fare un riferimento legato all'articolato della nostra Carta, fra l'articolo 32, che ho appena citato, e l'articolo 82 della Costituzione, che riconosce al Parlamento la facoltà, attribuendogli addirittura i poteri e i limiti della magistratura, di istituire delle Commissioni di inchiesta per acclarare ciò che ancora non è chiaro, per mettere in luce ciò che ancora è nell'ombra,

Non possiamo neppure immaginare che possa andare disperso il lavoro maturato fino alla scorsa legislatura, ma non possiamo neppure permetterci il lusso di pensare che i due anni contemplati dal documento per l'attività di questa Commissione possano o debbano addirittura essere ulteriormente prorogati, perché abbiamo la riserva mentale di trattare questa materia così delicata con una finta prudenza, dietro la quale si nasconde l'indisponibilità effettiva a cercare e a trovare la verità. Allora, collega Amato, in questa circostanza a lei e al sottosegretario Cossiga, per la parte importante e significativa che molto degnamente rappresenta, compete il compito di esprimervi in maniera esplicita ed inequivocabile. A proposito degli effettivi limiti che eventualmente si si dovessero imporre apertamente o in maniera surrettizia all'attività di questa Commissione, credo che un obiettivo liberatorio potremmo raggiungerlo mantenendo l'impegno assunto nel testo unificato a far attribuire la Presidenza di questa Commissione al Presidente del Senato.

Se si continua così, come se nulla fosse, ho due soluzioni: aumentare il volume o sospendere la seduta per un quarto d'ora. Regolatevi di conseguenza perché, se continua questo chiacchiericcio così diffuso e generalizzato,

la lunghezza del mio intervento sarà inversamente proporzionale all'attenzione che l'Aula mi riserverà.

Noi ci attendiamo dal Governo e dal relatore una risposta chiara sull'effettiva volontà di far funzionare questa Commissione sull'effettiva volontà di non accettare nessun tipo di limite e di condizionamento. Si parlava della Presidenza da far attribuire, com'è inserito nel testo originario, al Presidente del Senato. Il riconoscimento al Presidente del Senato di una potestà così importante e così delicata, a mio modesto modo di vedere, sottolinea la straordinarietà dell'evento. Immettere la nomina del Presidente in una fisiologia ordinaria, lasciando alla consistenza dei Gruppi il compito di decidere chi dovrà tenere il timone in mano, a mio giudizio, può voler dire che alla Commissione della XVI legislatura ne seguiranno molte altre, e intanto la verità non verrà acclarata, e intanto la giustizia non verrà fatta. concludo richiamando due elementi, perché è importante che almeno in questa occasione vengano sottolineati. Normalmente - questo accade soprattutto quando si individuano delle espressioni che vorrebbero poter rappresentare per intero il problema problema - si parla di sindrome dei Balcani, ma non basta, signor Presidente. Molti, infinitamente più autorevoli di me, sono convinti che ci sia la sindrome dell'Iraq, dell'Afghanistan e del Libano.

sarda, targata Sardegna, che potremmo definire sindrome del Salto di Quirra, sindrome di Escalaplano, sindrome di Perdasdefogu.

il cui livello di veridicità sfiora quello che, effettivamente, si vive là dove la guerra si E lì non muoiono soltanto i soldati (come se fosse poco vedere soldati che muoiono). Lì muore la gente; lì ci sono malattie diventate endemiche; lì si muore di leucemia

manifestando il mio voto convinto a favore dell'istituzione di questa Commissione e sottolineando, ancora una volta, quanto ho tentato di dire in apertura. Io mi fido dei colleghi che hanno lavorato a questa proposta. Io mi fido del senatore Amato, e mi fido del Presidente della mia Commissione, così come mi fido del sottosegretario Cossiga. Costoro dovranno dirci, prima della conclusione del dibattito, ancora una volta, che questa è l'occasione buona per dire la verità. Se così sarà, noi saremo i primi a batterci, con tutte le nostre forze, perché giustizia venga fatta.

Vorrei dire all'illustre collega che, da parte nostra, c'è tutta la volontà di non far fallire questa Commissione. Insieme, peraltro, noi abbiamo lavorato alla formulazione del testo della Commissione difesa e, insieme, abbiamo costruito un impianto. Nel costruire quell'impianto, abbiamo anche rivendicato una continuità con la precedente Commissione, la Commissione Menapace, e con quella ancora precedente, presieduta dal collega Franco perché è importante dare il senso di questa continuità. Nello stesso tempo, abbiamo introdotto delle novità per approfondire una questione

Quindi, una Commissione che vuole essere concreta nel suo operare. Certo, le garanzie di operatività sono date - comprendo il senso dell'intervento del collega Scanu - anche dall'assetto della Commissione.

oggetto della Commissione di inchiesta vi sia anche quella dell'esposizione di personale militare e civile al radon.

Casson e Balboni, perché hanno dato slancio ad una Commissione già prevista, che ha lavorato intensamente nelle due passate legislature e che adesso dovrebbe portare a buon fine, anche facendo tesoro di quello che è stato fatto in Alla luce delle vittime e delle malattie che hanno colpito i nostri concittadini incolpevoli e conseguentemente le loro famiglie, è veramente necessario fare definitivamente chiarezza e rendere giustizia al loro sacrificio e alle loro

il Presidente del Senato, ritengo che la Commissione sarà sicuramente in grado di esprimere un'onorevole Presidenza, anche perché, com'è stato poi sottolineato dallo stesso relatore Amato,

tra le patologie oggetto dell'inchiesta e singoli fattori di rischio all'esame delle indagini; tuttavia, data l'obiettiva sussistenza di fenomeni morbosi, anche con riferimento all'operatività di altre concause, si sono auspicati maggiori approfondimenti in merito, ed è questa la ragione per cui dobbiamo proseguire nel nostro lavoro. nostro lavoro. Dall'esame compiuto durante la scorsa legislatura, è emersa infatti la necessità di estendere il raggio di analisi ad un più ampio novero di fattori di rischio per la salute e alle loro possibili interazioni. Questo ulteriore approfondimento sarebbe funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di promuovere condizioni di maggiore sicurezza per il personale delle Forze armate e per la stessa popolazione civile e potrebbe servire a concorrere alla definizione delle responsabilità inerenti ai casi di morte e di gravi malattie verificatisi a carico di civili e militari, anche ai

ponendo l'onere della prova a carico dell'amministrazione. Emerge quindi dalla relazione redatta dalla precedente Commissione, la necessità di completare la raccolta e l'analisi epidemiologica e l'analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile interessato dall'oggetto dell'inchiesta, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale, sia di quello inviato nelle missioni internazionali all'estero, con particolare riguardo - cosa che riteniamo assolutamente opportuna e che ci trova particolarmente d'accordo - alla verifica degli attuali schemi di vaccinazione praticati e, soprattutto, delle modalità di preparazione degli stessi. Emerge pure l'urgenza di avviare un'indagine epidemiologica volta a verificare l'eventuale incremento del tasso di mortalità e delle malformazioni congenite nei bambini nati dal 1990 ad oggi dai militari

sia al fine di selezionare le migliori forme di sistemazione logistica ed i più opportuni equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate, sia al fine di garantire un continuo ed adeguato monitoraggio sui rischi di natura nucleare, batteriologica, chimica e radiologica, mediante la presenza costante di figure professionali specializzate e di attrezzature idonee. Riteniamo quindi necessario un approfondimento dei succitati aspetti, alla luce di una nostra ferma convinzione, che l'uranio impoverito non debba essere comunque utilizzato a fini bellici, stante la sua natura radioattiva e genotossica ed i sicuri effetti di inquinamento ambientale; è altresì necessario un approfondimento della ricerca sui suoi meccanismi di azione, soprattutto in relazione agli aspetti sinergici. Ciò che ci preme particolarmente è, inoltre, che la costituenda Commissione faccia luce sulle componenti e le modalità di somministrazione dei vaccini e sulle condizioni immunitarie dei soggetti destinatari, estendendo il raggio di indagine anche ai rischi associati alla presenza di gas radon e di materiale contenente amianto negli ambienti ove il personale militare presta servizio e, non ultimo, addivenendo alla definizione di una forma di indennizzo previdenziale e di sostegno al reddito per le famiglie. Riteniamo, infine, importante e condividiamo la decisione di far sì che la Commissione si proponga anche di monitorare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e, per quanto di competenza, della Sanità militare. La fruibilità dell'efficienza e l'efficacia di quest'ultima sul territorio italiano e all'estero è condizione primaria per assicurare la tutela della salute di tutti coloro che sono soggetti a rischio nell'espletamento del proprio servizio. Alla luce quindi dei troppi casi di morte e malattie che hanno colpito militari e civili incolpevoli di ritorno dalle missioni, è un dovere per le istituzioni cercare e trovare soluzioni, cercare e in modo che non si verifichino casi analoghi. Sarebbe a mio avviso opportuno tener conto e far tesoro dei pericoli che sono derivati dalle conseguenze dell'uranio impoverito anche per le scelte politiche che il Governo e questa Aula deve prendere in altri casi completamente diversi viene usato l'uranio e dove il problema delle scorie non è risolto, come, per esempio, nel caso dello sfruttamento dell'uranio per l'energia.

Presidente, colleghi, con grande leggerezza potremmo oggi semplicemente sostenere la proposta *bipartisan* di istituire una Commissione monocamerale d'inchiesta chiamata a indagare sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno. La sosterremo, ma la nostra coscienza, i nostri valori, l'impegno che abbiamo voluto assumere di fronte ai nostri elettori ci portano oggi a non limitarci a questo ma ad aprire un momento di riflessione di fronte a tale proposta. L'Italia dei Valori conosce il problema dovuto all'esposizione all'uranio impoverito ed è sensibile a tutte le richieste di aiuto che vengono dai dai militari che per anni hanno servito il nostro Paese all'estero e che ora si trovano ad affrontare un'altra sfida, quella più dura e difficile della malattia. Toccanti nuove vicende umane di persone che hanno contratto varie patologie dopo l'esposizione all'uranio impoverito sono purtroppo all'ordine del giorno ed il tema ha acquisito un'indiscussa attualità e urgentemente chiede una soluzione. Su questo punto, esimi colleghi, penso di poter affermare tranquillamente che siamo tutti concordi e che il pensiero sia univoco: lo testimonia questa proposta voluta fortemente sia dalla maggioranza sia da gran parte dell'opposizione. Non siamo però del tutto d'accordo sul modo in cui si intende dare risposta ai nostri militari, ai loro parenti ed all'opinione pubblica più in generale. colleghi, è giunto il momento di istituire una nuova - l'ennesima - Commissione d'inchiesta; per noi, invece, è sopraggiunta l'ora di passare ad una seconda fase, successiva e più incisiva. Siamo pronti a collaborare per la predisposizione di atti normativi che sappiano riconoscere i giusti diritti a chi è stato ed è vittima dell'esposizione a questi agenti patogeni. Noi riteniamo già di per sé accertati i danni ai soggetti che sono stati a contatto con l'uranio e ci auguriamo che sia lo stesso per voi. L'ultima Commissione cosiddetta sull'uranio impoverito, che ha visto la luce l'11 ottobre 2006, era composta da 21 senatori ed ha effettuato complessivamente 13 sedute in sede plenaria, 20 riunioni dell'ufficio di Presidenza (allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari), una missione in provincia di Lecce, nonché due sopralluoghi in Sardegna e uno in Libano. Un'agenda fitta, dunque, di impegni, di dibattiti e di audizioni di prestigiosi e autorevoli collaboratori. Sono stati sentiti, infatti, i rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità nelle sedute dell'11 e del 17 aprile 2007, e della Direzione generale della Sanità militare, il 17 maggio dello stesso anno: esperti qualificati e scienziati che da anni studiano il problema. Il serio e notevole lavoro svolto dalla Commissione in questione ha portato alla realizzazione di una importante relazione finale. La Commissione d'inchiesta appena citata ha portato avanti infatti i lavori già iniziati nella XIV legislatura ampliandoli e integrando i dati precedentemente raccolti. Non ci si è limitati ad una mera verifica degli effetti dall'esposizione all'uranio impoverito per le Forze armate, ma sono stati presi in considerazione altri possibili fattori di rischio rischio che potrebbero avere innescato le patologie che oggi presentano i militari e le popolazioni civili residenti nei territori dilaniati dai conflitti. Nel corso dei lavori è emersa la necessità di disporre di dati più completi ed accurati, e a tal fine si è giunti a promuovere un'attività sistematica di raccolta dei dati presso i competenti uffici del Ministero della difesa, mediante la formulazione di quesiti volti ad individuare il personale militare ammalato o deceduto nel decennio Sebbene a conclusione dei lavori di raccolta dati sia emersa la necessità di avviare un'indagine più scrupolosa e che abbia a disposizione più tempo, il lavoro svolto è stato giudicato dalla Commissione - cito testualmente - «interessante». Bene, colleghi, tra i nuovi compiti che il documento in esame intende affidare alla Commissione di questa legislatura rientra, all'articolo 1, comma 1, lettera c*)*, quello di valutare l'«adeguatezza della raccolta e della analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero». Mi auguro che così facendo non si metta in dubbio quello che la precedente Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito ha definito un interessante lavoro e non ci si arroghi, quindi, la presunzione di stabilire che in soli tre anni le metodologie di raccolta dati siano migliorate notevolmente tanto da giustificare l'avvio di una nuova ricerca, con tutti i costi che questa comporta. La nostra speranza è che da quella ricerca si proceda e si vada avanti e non se ne annullino i risultati. Io non credo, e mai lo affermerò, che il nostro agire possa essere indipendente e non debba tener conto dei fatti reali, ma sono convinto che, almeno in questo caso, non possiamo permetterci di perdere altro tempo e attendere ancora che gli studi diano Come, correttamente, è stato sostenuto dall'ultima Commissione d'inchiesta, è giunto il momento di abbandonare l'ipotesi di poter stabilire, con dati certi, un possibile legame tra le patologie oggetto dell'inchiesta e l'esposizione all'uranio impoverito o ad altri agenti nocivi, e introdurre il cosiddetto criterio di probabilità quale riconoscimento sufficiente per poter avere accesso agli strumenti risarcitori. In seno alla scorsa Commissione d'inchiesta, una folta schiera di consulenti ed esperti ha chiaramente segnalato la natura genotossica dell'uranio impoverito, e già nel 2000 la cosiddetta commissione Mandelli aveva appurato come, in seguito alla guerra dei Balcani, il numero di militari vittime di linfomi di Hodgkin Colleghi, quale altra conferma attendiamo? Perché oltre ad autorizzare ed istituire una nuova Commissione d'inchiesta non procediamo al vaglio di una seria e dettagliata normativa che sappia garantire i diritti che oggettivamente dovrebbero spettare ai nostri soldati? Un'altra criticità: tra i compiti che questa Assemblea intende affidare alla futura Commissione rientra quello di indagare, come sancito all'articolo 1, comma 1, lettera b*)* «sulle specifiche condizioni ambientali dei vari contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate». La Commissione sull'uranio impoverito questo importante lavoro di accertamento e valutazione lo ha già svolto, colleghi, ed ha già reputato fondamentale proteggere adeguatamente i soldati inviati in zone di guerra, sia sotto l'aspetto logistico che dal punto di vista dell'equipaggiamento.

non vale la pena correggere le troppe ed eccessive enfatizzazioni ed imprecisioni che sono state fatte fino adesso. Da più di cinque anni si è lavorato, con più Commissioni, per cercare di trovare un nesso di causalità tra esposizione e rischi. Signori miei, non ci siamo riusciti, ma non è detto che non ci si possa riuscire. Quello che noi vorremmo, che abbiamo voluto e che continuiamo a volere è trovare le ragioni perché i malati e le famiglie possano avere un giusto riconoscimento, un risarcimento dei danni o comunque un ristoro economico. Da quanto è emerso fino adesso, la radioattività dell'uranio impoverito è praticamente nulla. L'unico dato emerso è che soltanto lo scoppio

però restringere l'area del risarcimento a quei pochi militari che si sono trovati nei teatri di guerra, anzi sui fronti di guerra. Premesso ciò, con tutte le perplessità che abbiamo sull'argomento, vorremmo dare ancora una speranza alle famiglie, per cui siamo favorevoli all'istituzione di una

Non stiamo facendo archeologia di un'indagine, ma stiamo cercando verità e giustizia, perché continuano a giungere anche oggi, da ogni parte del Paese, segnalazioni di patologie di vario genere che hanno colpito militari italiani, in Italia e all'estero. Per questo motivo, esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta che, come Partito Democratico, abbiamo richiesto e auspicato fin dall'inizio della XVI legislatura, ormai circa due anni fa. A questa nostra richiesta, qualche mese dopo si è associata una proposta del PdL, di cui è stato il senatore Balboni, che conteneva delle richieste molto simili, specialmente relativamente alle finalità, oltre ad aspetti che sono stati integrati dal lavoro della Commissione. Va detto in via preliminare che questa Commissione non va intesa come atto critico nei confronti delle Forze armate o come contrapposizione al lavoro che queste svolgono. Essa muove queste svolgono. Essa muove dall'obiettiva necessità di approfondire diversi profili relativi al rischio sanitario del personale militare, secondo le indicazioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nella scorsa legislatura e anche nella XIV. In particolare, In particolare, si impone uno strumento di inchiesta perché le singole indagini della magistratura su tali temi non sono mai riuscite a dare risposte certe e definitive. Nel frattempo, va detto che il lavoro svolto dalla Commissione difesa è stato proficuo, tanto da giungere alla comune convinzione della necessità di estendere l'oggetto dell'inchiesta, anche in base alle sollecitazioni giunte da singoli cittadini militari, nonché da organizzazioni ed associazioni che curano gli aspetti più delicati dell'intera questione. È così che, oltre ad occuparsi di uranio impoverito e di nanoparticelle, la Commissione istituenda dovrà anche indagare sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego, dovrà indagare sulle modalità della somministrazione dei vaccini allo stesso personale, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, dovrà indagare sui rischi associati alla presenza di gas radon o di materiali contenenti amianto negli ambienti dove il personale militare è chiamato a prestare servizio. La recente vicenda del processo instaurato a Padova nei confronti di alcuni vertici militari per il decesso di militari della Marina militare e le indagini partite per circa altre 600 vittime militari da amianto danno contezza della necessità di questo approfondimento. Infine, bisognerà indagare sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito, attualmente previsti dall'ordinamento a favore dei soggetti colpiti da patologie correlate. il compito cui è chiamata la Commissione è estremamente vasto, gravoso e molto impegnativo. È peraltro foriero di buoni risultati il fatto che si giunga oggi ad un voto favorevole condiviso da tutti, perché tutti ci rendiamo ben conto della necessità di tutela dei nostri militari, dei lavoratori militari, colpevoli solo di aver fatto il proprio dovere, a seguito del quale risultano essersi ammalati e in certuni casi risultano deceduti per gravi patologie tumorali. Ma il valore principale di questa nostra decisione favorevole consiste nel riconoscere l'imprescindibilità istituzionale delle esigenze di verità, di tutela, di giustizia, di solidarietà. Vogliamo sapere che cosa è successo; vogliamo sapere per quale motivo i nostri militari si sono ammalati o sono deceduti: vogliamo saperlo anche per tutelare e salvaguardare coloro che ancora stanno affrontando analoghi scenari di guerra, o che in Italia stanno svolgendo attività collegate. Vogliamo rendere giustizia ai nostri morti, vogliamo concretamente, come istituzioni, essere vicini alle vittime, in uno spirito di solidarietà che caratterizza parti fondamentali della nostra Costituzione. È un dovere che abbiamo nei confronti di tutte le vittime, sia militari che civili, e nei confronti dei loro familiari; è un dovere etico, sociale, politico al quale il Parlamento non si può sottrarre. *(PdL)*. Signor Presidente, il Popolo della Libertà voterà a favore dell'istituzione della Commissione di inchiesta perché ritiene che sia l'adempimento di un dovere morale nei confronti delle migliaia di giovani che si sono ammalati di gravi e gravissime malattie degenerative, tra l'altro tipiche non della giovane età ma di una popolazione in età avanzata, delle centinaia di militari che sono morti, dei loro familiari, di tutti coloro che hanno sofferto. È giusto proseguire nell'indagine, perché le precedenti Commissioni, pur con un lavoro encomiabile, non hanno raggiunto una certezza definitiva. Vi sono elementi che fanno ritenere che oltre o al posto di un fattore patogeno come l'uranio impoverito vi possano essere altri fattori, in particolare i vaccini e la loro modalità di somministrazione, e i protocolli con cui venivano somministrati. Ci sono tanti giovani che non sono mai stati all'estero, che non sono mai stati sui teatri nei quali è stato impiegato l'uranio impoverito e che ugualmente si sono ammalati, e molti di questi sono morti. Quindi, con tutto il rispetto delle conclusioni precedenti, noi riteniamo che bisogna approfondire, allargare l'indagine, acquisire ulteriori dati, perché prima di tutto occorre raggiungere la verità, occorre dare risposte ai familiari e al Paese, perché questi giovani che credevano nella Patria, che credevano nei nostri stessi valori, hanno perso la vita, e ciò non si deve più ripetere. Questo è anche l'unico modo per rendere giustizia e per avviare quei giusti risarcimenti che certamente i familiari e gli ammalati si aspettano. Per questo motivo noi votiamo a favore dell'istituzione di detta Commissione

*(PD)*. Signor Presidente, mi si consenta di segnalare e illustrare brevissimamente la drammatica situazione di un folto nucleo di ex lavoratori della pomice nell'isola di Lipari che, disoccupati, dimenticati e abbandonati negli ultimi tre anni dalle autorità locali, regionali e nazionali, occupano da quindici giorni l'ufficio del sindaco nel capoluogo eoliano, effettuando al contempo uno sciopero della fame, causa del ricovero in ospedale di 6 di loro in preoccupanti condizioni. Il gruppo di questi 40 disperati costituisce solo una parte di oltre un centinaio di ex dipendenti licenziati dalla società pomicifera Pumex, che cessò le attività nel dicembre del 2006. Gli operai di quella che era stata da sempre la più importante azienda e fonte di lavoro dell'arcipelago eoliano hanno visto svanire ogni speranza legata alle promesse ed agli impegni, mai mantenuti, del Ministero dei beni culturali,

cave di pomice e riconversione del territorio in Parco geominerario, con opere finalizzate ad un turismo culturale e naturalistico.

Si tratta di una questione che riguarda un territorio a scavalco fra la Regione Veneto e la Regione Lombardia. Premetto che mi rendo conto della competenza e del fatto che si tratti di un territorio così importante che non sfugge all'attenzione del Governo. Credo, però, che non debba sfuggire soprattutto ad un membro del Governo che si candida ad essere Presidente di questa importante Regione del Nord-Est. Scavalcando tutti i piani territoriali generali dei Comuni confinanti, Provincia di Verona e Provincia di Mantova, la Regione Veneto ha dato la concessione per la costruzione del più grande centro commerciale d'Europa con l'illusione, anzi con lo specchietto delle allodole della costruzione di una *motor city*. Le piste per le automobili o per le moto sembrano ormai diventate un miraggio per tutti i nostri territori, quasi si tratti di strumenti di valorizzazione e sviluppo. Purtroppo la la concentrazione di PM 10 e di traffico in quella zona diventerà insopportabile. Avremo poi conseguenze di carattere sanitario e forse conseguenze *ex post* - ahimè

Molti elettori vogliono sapere, con insistenza, quanti e quali soldini pubblici hanno percepito e stanno percependo, a vario titolo, le associazioni ambientaliste, animaliste, anticaccia, antitutto praticamente,

e con quali costi a carico dei cittadini. Spesso si vuol far passare il cacciatore come un bracconiere, ma tutti noi sappiamo che non è così. Per quanto riguarda le Per quanto riguarda le accuse di presunto maltrattamento di animali, nonostante l'archiviazione dei procedimenti, gli animali sequestrati non sono mai stati restituiti ai legittimi proprietari. Non vorrei sussistesse un manifesto interesse, anche di natura economica, da parte delle associazioni alle quali vengono affidati questi animali posti sotto sequestro a far durare il più lungo possibile i tempi di custodia degli stessi. Chiedo, inoltre, nella mia ultima interrogazione, di sapere quali sono i criteri di valutazione adottati per rendere tutte queste associazioni - quelle che ho citato prima e le altre - delle ONLUS che, con tutti i vantaggi economici che ne derivano, continuano a diffondere messaggi menzogneri con allarmismi che, di fatto, non esistono. Signor Presidente, ancora una volta chiedo di porre all'attenzione di quest'Assemblea la vertenza dei lavoratori della Fincantieri di Palermo. Oggi le rappresentanze sindacali hanno diffidato l'azienda a non attuare la proroga della cassa integrazione guadagni (CIG) perché esistono le condizioni per occupare i lavoratori.

un chiaro segnale positivo ai lavoratori palermitani. Nel contempo sollecito ancora una volta il ministro Scajola affinché dia avvio alle commesse pubbliche promesse a settembre 2009 ed intanto lo invito a incontrare le rappresentanze sindacali visto che l'8 marzo l'appuntamento è stato disdetto. Inoltre, a dimostrazione che la crisi non è psicologica, vorrei evidenziare, così come ha fatto il collega Randazzo, la grave situazione dei lavoratori della ex Pumex che nelle isole Eolie hanno avviato uno sciopero della fame, Dopo che nel 2000 l'area ha avuto il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, non è stata ancora avviata la riconversione dell'area di estrazione della pomice a Lipari; nonostante le promesse del governo regionale allora in carica e ora del Governo nazionale non si è visto alcun impegno concreto. Chiedo pertanto che la Presidenza avvii l'iniziativa necessaria per dare un concreto impulso all'attività del Governo nazionale.

*(PD)*. Signor Presidente, purtroppo mi trovo a richiamare un ordine del giorno che è stato adottato un anno fa in quest'Aula relativamente alla ratifica del Trattato Italia-Libia

in Parlamento, arricchire il rapporto con il dittatore Gheddafi e, da tre settimane a questa parte, aprire un contenzioso diplomatico con la Svizzera. pare che il ministro Frattini ieri si sia recato a Tripoli per creare qualcosa come un regolamento speciale per consentire ai 186 libici sulla lista nera preparata da Berna di entrare comunque nella zona Schengen e tra questi naturalmente c'è anche Gheddafi. Tra i temi che dovremmo discutere nelle Aule parlamentari probabilmente, più di ciò che è già stato ratificato con un Trattato, ci dovrebbero essere i motivi per cui si decide di rompere con un alleato storico e nostro vicino come la Svizzera per andare invece incontro alle esigenze di un dittatore.

di mezzo milione di euro a fronte dei cinque miliardi che daremo alla Libia. Non è mai stata data una risposta esauriente alla domanda

questa distrazione di fondi. Si tratta di 20 miliardi di euro sottratti ai progetti per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate e adoperati per tutt'altro: l'ultima, ma non ultima, la puntuale analisi corredata di cifre e riferimenti dell'onorevole Tino Iannuzzi. Sui fondi FAS vogliamo chiarezza e verità. Il Governo venga in Aula a spiegare al Parlamento e al Paese perché questi fondi sono stati sottratti a quelle aree. Signor Presidente,

Signor Presidente, mi rivolgo a lei e alla Presidenza del Senato per chiedere di assumere una tempestiva iniziativa presso il Governo in ordine ad una questione molto delicata che ho già sottoposto per iscritto alla valutazione e considerazione del signor Ministro dell'interno. Mi riferisco alla necessità assoluta di una tempestiva modifica della pubblicità elettorale istituzionale che da alcune settimane è in diffusione sulle reti televisive nazionali. L'illustrazione del sistema di voto, signor Presidente, è riferita in massima parte alle Regioni italiane interessate al prossimo turno elettorale nelle quali, però, vigono determinate norme in materia, per l'appunto, elettorale. Si parla, infatti, di listino, listino, di preferenza unica e soltanto alla fine del messaggio pubblicitario si fa riferimento a cinque Regioni (la Toscana, le Marche, la Campania, la Puglia e la Calabria) in cui il sistema elettorale

genere. Credo che questo fatto vada spiegato al corpo elettorale. Esprimo la preoccupazione che la diffusione di un messaggio così fuorviante possa disorientare buona parte del corpo elettorale. È necessario dunque che si assuma subito un'iniziativa, data la prossimità della consultazione elettorale, magari facendo in modo che le reti televisive (almeno la RAI in sede regionale) possano diffondere messaggi più mirati e appropriati e appropriati non disorientando l'elettorato e mettendo tutti in condizione di esprimere correttamente il proprio consenso sulla base di valutazioni e di informazioni certe ed attendibili. *(Applausi della Signor Presidente, intervengo per segnalare all'Aula e alla Presidenza la situazione di grave disagio che si è venuta a creare in Provincia di Milano per la chiusura inopinata e ingiustificata delle alzaie del Naviglio grande. grande. A fronte di una sentenza alquanto discutibile che ha disposto un risarcimento in capo al Parco del Ticino, lo stesso ha deciso di chiudere la pista ciclabile che passa lungo le alzaie del Naviglio, fatta da Leonardo qualche anno fa. È di tutta evidenza che è impossibile pensare che sulle alzaie del Naviglio si possano mettere *guard rail* o qualcosa di simile; la soluzione andrà trovata in altro modo. Quello che volevamo segnalare, cosa alquanto interessante, è come a fronte di una scelta così sbagliata la popolazione abbia reagito nel migliore dei modi, e cioè

L'interrogazione faceva riferimento ad una precisa denuncia del revisore dei conti della Metro Roma, il dottor Simplicio Di Caterino, che denunciava questo obbrobrio e e bloccava il pagamento di questo appannaggio al dottor Monorchio, che poi è stato rierogato anche se non si sa per quale motivo. al Ministro delle infrastrutture se rientravano queste cifre nei costi specifici per i collaudi dell'azienda della metropolitana o di qualsiasi azienda di trasporto pubblico della nostra Regione. Anche se spa, queste nomine sono concordate tecnicamente con gli uffici dei competenti Ministeri. Quindi, data l'importanza e data la situazione economica del Paese e, in particolare, anche quella della città di Roma, io ritengo che questa interrogazione debba avere la sua attenzione, affinché lei possa sollecitare il Governo ad una risposta che, anche se tardiva, è sicuramente importante.